Signor Presidente, signor Ministro dello sviluppo economico, onorevoli colleghi,

che ha determinato la fuoriuscita di gas radioattivi dalla centrale nucleare di Fukushima,

assunto una posizione, condivisibile, di sospensione del piano nucleare, demandando ad una verifica delle condizioni di sicurezza. L'emendamento presentato ieri sera, però, pone in modo molto più netto e deciso il problema dell'abrogazione del piano nucleare, riattivato da poco tempo per il nostro Paese. È su questo che vorrei attirare, se è possibile, l'attenzione dei colleghi e del Governo. Quali sono le conseguenze economico‑sociali di questa decisione, a fronte delle quali, ovviamente, devono esserci sacrosante valutazioni dei rischi che un piano nucleare può comportare? Queste conseguenze, anche se in modo un po' approssimato, possono essere basate su dati storici. Basta riferirsi alla precedente decisione che, sull'ondata emotiva di Chernobyl, portò al *referendum* e, quindi, a quella che erroneamente è stata definita l'uscita dell'Italia dal nucleare. Qui, cari colleghi, occorre fare chiarezza: l'Italia non è mai uscita dal nucleare, né mai uscirà dal nucleare. Quella decisione ha comportato l'uscita dell'Italia dalla produzione di energia nucleare, ma la permanenza del nostro Paese nel consumo di energia nucleare. nucleare. Se facciamo i conti, negli ultimi 20 anni, il maggior prezzo dell'energia elettrica è stato pagato da ogni famiglia italiana,

di far uscire l'Italia dalla produzione di energia nucleare, ma di rimanere nel consumo dell'energia nucleare, con la conseguenza che l'abbiamo comprata all'estero,

costi. Quel maggior costo di energia elettrica corrisponde, cari colleghi, a 21 centrali nucleari. In questi 21 anni, gli italiani hanno, pagando di più l'energia elettrica, pagato 21 centrali nucleari francesi. un terzo delle 62 centrali nucleari francesi è stato pagato dai consumatori italiani. Se questo è il dato storico, la decisione...

Questi sono i dati storici, questo è quanto è avvenuto. Noi italiani dovremmo oggi essere proprietari di un terzo delle centrali nucleari francesi: non ne abbiamo la proprietà, ma ne abbiamo pagato il costo. il costo. Se questo è il dato storico, se proiettiamo la decisione che ci viene proposta oggi sui prossimi venti anni, fra venti anni l'Italia avrà pagato 42 centrali nucleari francesi, e fra venti anni ancora avrà pagato l'intero parco delle centrali nucleari francesi (62 centrali), attraverso

di un basso prezzo dell'energia elettrica, mentre l'alto costo degli investimenti e degli impianti sarà stato pagato dai consumatori italiani.

Mi permetto di far osservare che sono personalmente estremamente favorevole alle fonti rinnovabili, che hanno bisogno però di ricerca e di innovazione, perché, allo stato attuale della conoscenza tecnico‑scientifica, le fonti rinnovabili, in realtà, rischiano di rinnovare le truffe vissute in tutti questi anni. Mi riferisco, ad esempio, al caso del fotovoltaico, dove il consumatore italiano, che già paga l'energia elettrica di più per pagare le centrali francesi, di più per pagare le centrali francesi, paga di più l'energia elettrica anche per dare un sussidio

per cento che va direttamente nei ricavi, puliti e netti, dei conti economici di coloro che fanno questo tipo di investimento. Questi soggetti operano in piena legittimità, perché è una legge che consente loro di usufruire di questo tipo di incentivo. Quindi, giustamente, se la legge lo consente, è opportuno che gli operatori più intelligenti e più avveduti lo utilizzino. Allora mi chiedo, ministro Romani,

e rivolgo una richiesta formale in quest'Aula, signor Presidente, in relazione all'altro provvedimento, al Documento di economia e finanza. In questo mi rivolgo al Ministero dell'economia e delle finanze,

che l'abrogazione del piano nucleare cambia radicalmente i numeri del Documento di economia e finanza, quello che dovremmo discutere a partire dal prossimo 3 maggio. Allora, chiedo formalmente che sia prevista una nota integrativa, possibilmente entro la prossima settimana, al Documento di economia e finanza, per capire come gli investimenti sul nucleare e i costi dell'energia impattano in quei documenti che oggi diventano numeri fragili ed incerti, ma certamente non adatti ad un serio confronto parlamentare. Se dovessimo discutere delle tabelle disponibili ad oggi (D, E e F), discuteremmo avendo incorporato il piano nucleare, quel piano nucleare che non c'è più. Chiedo allora una nota integrativa che aggiusti il quadro

ha adottato un decreto-legge con il quale si dispone la sospensione dell'efficacia del decreto legislativo n. 31 del 2010, e ha dovuto fare questo condizionato dalle decisioni assunte in sede comunitaria. Ieri pomeriggio ci è stato consegnato un emendamento che prevede, a differenza del testo del decreto-legge, non più la sospensione dell'efficacia, bensì l'abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari. Il Ministro sostiene che l'emendamento è la naturale conseguenza della sospensione dell'efficacia. Questo è un mistero, Ministro. Se avesse modo di potercelo spiegare, gliene saremmo grati. Afferma anche che questa decisione è perfettamente coerente con la strategia energetica, di cui non vi è traccia negli atti conosciuti assunti dal Governo o sottoposti al vaglio del Parlamento. Ci comunica inoltre che, sulle rinnovabili, occorre insistere ed investire, magari agendo in coerenza con il testo del decreto legislativo sulle rinnovabili, varato nel disprezzo più totale del parere reso all'unanimità da Camera e Senato, con il quale invece sono stati bloccati tutti gli investimenti sulle rinnovabili; provvedimento tanto discusso da indurre il Governo ad annunciare un nuovo provvedimento, da assumere in tempi estremamente veloci, per correggere quello appena varato. Anche di questo provvedimento non conosciamo ancora il testo. Solo qualche settimana fa il ministro Tremonti rassicura il Paese, preoccupato per la scarsa o nulla capacità di reazione alla crisi, mentre gli europei - come sappiamo - hanno ripreso a crescere anche in maniera significativa: Tremonti annuncia che con il nucleare il PIL crescerà molto di più. Qualche ora fa lo stesso Ministro, in Commissione bilancio, di ritorno da Bruxelles ove ha avuto modo di esprimere le proprie valutazioni, ci ha confortato segnalando come sia un bene per l'Italia non avviare il nucleare per gli alti costi di investimento e di gestione necessari e per i costi non stimati e non stimabili per la gestione in sicurezza dei rifiuti. In Italia - dice ancora il Ministro - non dobbiamo sostenere i costi per le bonifiche dei siti radioattivi, cosa che devono fare altri Paesi europei. Quindi siamo avvantaggiati e possiamo investire sulle rinnovabili, sul cui sviluppo deve impegnarsi tutta l'Europa. l'Europa. A fine anno 2010 - quindi solo poche settimane fa - nel programma nazionale delle riforme, approvato e proposto dal Governo, si è assunto che il nucleare costituisse una componente essenziale per il futuro dell'Italia e, per questo, da realizzare subito. Il nucleare - si dice - è l'unica fonte in grado di garantire la crescita dell'economia italiana. Signor Ministro, qual è la posizione del Governo italiano? Qual è la strategia energetica e come si pensa di sostenere lo sviluppo industriale del nostro Paese? Quale ruolo giochiamo in Europa?

trucco per fermare i quesiti referendari». Altro titolo: «Il *blitz* deciso dopo un sondaggio e la paura di favorire il *quorum*». Altro titolo ancora: «Cancellato un programma nato male». Ancora: «Un Paese senza politica energetica». Ancora: «Centrali nucleari: abbiamo scherzato».

dalle dinamiche e delle iniziative proprie dei Paesi più avanzati, che in Europa stanno costruendo una risposta alla crisi e stanno agendo per cavalcare la ripresa che comunque ci sarà. In Italia, invece, è da tre anni che l'incertezza e la confusione regnano sovrane. Si blocca immediatamente il progetto strategico Industria 2015 perché varato dal precedente Governo, salvo poi annunciare di volerlo riprendere quando ormai erano state vanificate significative potenzialità. Si blocca il credito di imposta del 55 per cento sull'efficienza energetica, che aveva generato uno straordinario impegno di investimenti da parte dei privati, di avvio di nuove imprese, di creazione di nuova occupazione e di ingegnerizzazione di tecnologie mature e impiegabili in condizioni di sostenibilità su vasta scala. Si blocca un processo virtuoso che era stato avviato, salvo poi disporne la ripresa con tempi di ritorno del credito di imposta non più praticabili e significativi per le decisioni che i cittadini italiani assumono. Sulle rinnovabili si fa una cosa e se ne aggiunge un'altra. Sull'energia elettrica e sul gas si rallentano i processi di liberalizzazione a danno dei cittadini e delle imprese; si aumentano le accise sui carburanti, tanto da far lievitare i prezzi a livelli insostenibili. Non si fa nulla, signor Ministro, nonostante gli orientamenti assunti dal Consiglio d'Europa, per potenziare le reti di trasmissione e di interconnessione con l'Europa. Gli imprenditori sanno bene che, se si potesse comprare energia sul mercato europeo, il costo diventerebbe equiparabile a quello più basso praticato in quei Paesi. Signor Ministro, noi pensiamo che sia doveroso per gli interessi del Paese definire una linea se ciò non vi sembra contrario agli interessi del Paese, definite una linea valorizzando le competenze tecnico-scientifiche del nostro Paese, le capacità realizzative e imprenditive presenti, sviluppando - se possibile, signor Ministro - un rigore programmatico minimo. Sappiamo che siamo alla fine della legislatura, ma l'Italia non merita altri danni. Signor Ministro, occorre evitare nuovi pasticci. Infine, si valorizzi il lavoro del Parlamento. La 10ª Commissione del Senato ha avviato da mesi un lavoro per contribuire a definire la strategia energetica del nostro Paese. Signor Ministro, guardi agli interessi reali del Paese. In ultimo, vorrei aggiungere che per i settori esclusi dai provvedimenti citati (gli impianti di stoccaggio dei rifiuti, gli impianti per l'arricchimento del combustibile nucleare o per le attività di *decommissioning)* valgono le stesse problematiche di sicurezza. I sani principi di precauzione vorrebbero che anche quegli impianti vengano sospesi in attesa di norme più congruenti, aspettiamo un incidente che magari può verificarsi in qualche parte del mondo in riferimento a quegli impianti?

Il Popolo della Libertà prende atto della scelta del Governo poc'anzi esposta dal ministro Romani e presentata qui al Parlamento con l'emendamento 5.800

È una decisione difficile, perché il Governo nel 2008 ha avuto il coraggio di ripresentare l'opzione nucleare al nostro Paese; ha avuto questo coraggio e ha implementato la decisione del 2008 con varie iniziative legislative. Ora, con saggezza, con senso di responsabilità di fronte agli interessi del Paese, decide di chiudere, ed è una chiusura - ripeto - senza appello per quanto riguarda questa legislatura. personale amarezza. Sono un ingegnere nucleare che ha svolto per 27 anni questo lavoro e sono convinto della bontà di questa tecnologia. Devo però assolutamente condividere,

come dagli incidenti. Dopo il grave incidente di Three Mile Island del 1979, vi è stata una rivoluzione nella progettazione dei reattori nucleari per assicurare

perché l'incidente di Fukushima sia elaborato, metabolizzato, introdotto negli standard di sicurezza - come ha detto il ministro Romani - e nelle progettazioni. Non dimentichiamo che in Europa,

quindi una piena coerenza tra la chiusura del nucleare per questa legislatura e il subentro di una nuova Strategia energetica elaborata entro 12 mesi. In conclusione, tutti questi elementi mi confortano nel rassicurare

Presidente, siamo molto soddisfatti del *de profundis* che si sta recitando da ieri sull'avventura nucleare nella quale il Governo Berlusconi voleva imbarcare il nostro Paese fin dall'inizio della legislatura. Parlo di *de profundis* perché riconosco all'onestà intellettuale di un nuclearista convinto come il senatore Possa

non c'è che la fuoriuscita dal nucleare per i Paesi che avevano imboccato questa strada nei decenni scorsi. Infatti, la Germania ha avviato concretamente l'uscita dal nucleare, e sarebbe stato ben curioso che un Paese come l'Italia, che ha la fortuna di non avere centrali nucleari sul proprio territorio, ci si imbarcasse proprio adesso. Quindi, quella che stiamo celebrando in queste ore qui al Senato però al Ministro e ai colleghi della maggioranza: questa chiusura è amaramente condita da un eccesso di furbizia da parte vostra. Il ministro Romani ha ricostruito i giorni immediatamente successivi all'incidente di Fukushima. *(Brusìo).* Presidente, posso chiederle un aiuto?

continuare ad insistere era impossibile. Dispiace che ancora adesso, in queste ore, una persona autorevolissima, che è stato nostro collega fino a pochi giorni fa ed al quale tutti noi dobbiamo gratitudine per il lavoro che l'ex senatore Veronesi, oggi Presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, invece di tutelare il suo ruolo terzo come dovrebbe fare chi presiede quell'agenzia, continui a spingere su una scelta tecnologica che la storia si è incaricata di indicare come obsoleta.

un emendamento che ha l'unico obiettivo concreto di non far celebrare il *referendum* dell'11 e 12 giugno, mantenendovi poi aperte le possibilità di localizzazione del deposito secondo procedure che non sono affatto rispettose del consenso locale e riservandovi un diritto di

perché bisogna, una volta per tutte, affrontare i problemi che riguardano l'approvvigionamento, la diversificazione delle fonti, l'alto costo dell'energia per le piccole e medie imprese,

(sia con il lavoro della Commissione dei primi di marzo, sia con la risoluzione del Consiglio europeo), non fa altro che definire,

approvare un nuovo quadro normativo e regolamentare che i Paesi europei saranno obbligati a recepire attraverso una direttiva. Sia chiaro il *mix* energetico rientra nella sovranità di ogni singolo Stato membro ed è qui che non dovete giocare con l'equivoco e per questo abbiamo parlato

nella sua relazione, signor Ministro, ci sono due affermazioni molto gravi. La prima è che la scelta del Governo di non procedere è dettata - sono sue testuali parole - «dal fatto che non vi sono elementi di sicurezza». Signor Ministro, la sua affermazione è molto grave, perché dall'inizio della legislatura questo Governo ha varato ben tre provvedimenti legislativi in cui ha definito e riconfermato la scelta del nucleare. Lei, a distanza di tre anni, viene a dirci, dopo la scelta

tutto ha fatto tranne che scegliere il confronto. Infatti, la politica nucleare della localizzazione e costruzione delle centrali nucleari, secondo i provvedimenti di legge che avete approvato, potrà essere fatta contro la volontà delle Regioni, contro la volontà dei Comuni e contro la volontà dei cittadini. Ora, a distanza di tre anni, ci viene a parlare di confronto. Per tale ragione chiediamo che questo emendamento e il subemendamento vengano presi nella dovuta considerazione.

Presidente, innanzitutto voglio ringraziarla per l'opportunità che mi ha dato di intervenire ora, non avendolo potuto fare prima.

Non più di qualche settimana fa ci siamo trovati in questa Aula - lei presente - a discutere di mozioni che riguardavano appunto le energie rinnovabili e tutti i problemi connessi ad un piano energetico nazionale che doveva vedere il Governo presentare un paniere presentare un paniere di offerta di energia diversificato, perché il nostro Paese, che ha un così grande debito energetico ed è costretto ad importare e a pagare l'energia delle centrali nucleari francesi, ad ad importare il gas dalla Libia e dalla Russia, ha bisogno di una politica energetica che deve essere l'asse strategico del Governo.

per quali motivazioni c'è stato questo cambiamento rispetto ad una moratoria che avevamo accettato in quanto, per una certa sensibilità sia sociale che culturale, c'era un impegno morale e politico a fare una riflessione dopo quanto era avvenuto a Fukushima, che ovviamente doveva impegnare anche il Governo italiano, ancorché la politica energetica nel settore del nucleare fosse stata delineata e il Piano energetico nazionale fosse stato già votato e deliberato. Quindi, mi sono chiesta perché. L'unica spiegazione convincente che mi sono data è che comunque il Governo stia portando avanti una politica strabica, perché da una parte è attento

tutto quello che possiamo e vogliamo dire, perché ognuno ha diritto alla sua posizione. Io sono esponente di un partito che non è mai stato contro il nucleare, anzi ha fatto delle battaglie *pro* nucleare, perché condivide una politica che guardi alla scienza, alla tecnologia e allo sviluppo senza paraocchi, senza freni inibitori che non sono

rispetto a quel che andava dicendo da tutte le parti fino a qualche tempo fa. Per questo siamo profondamente delusi. Avremmo voluto che, al di là di quello che oggi è stato deciso, ci fosse comunque anche la sensibilità per poter dire a quest'Assemblea e al Paese che la scienza non si ferma, che le ricerca sul piano nucleare va avanti, perché è là che si dovranno trovare le prospettive per una energia pulita,

di cui non parliamo quasi mai. Non è soltanto una questione delle centrali nucleari. È una questione molto più complessa, che dovremmo guardare con la lente di ingrandimento, facendo attenzione alla sicurezza, facendo attenzione che non ci siano speculazioni nazionali e internazionali o di parte, facendo attenzione che prevalga la scienza per quello che è, con la capacità dell'essere umano di guardare ad essa con fiducia, scommettendo anche sullo sviluppo scientifico e tecnologico in questo Paese, che è sempre stato una Cenerentola. Pensiamo soltanto a cosa è successo al nostro Istituto nazionale di fisica nucleare, che ha visto partire i migliori cervelli,

l'abrogazione di tutta la normativa concernente il programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti nucleari. Si tratta di una normativa che, fra l'altro, era stata individuata nell'ambito del quesito referendario. Confermo pertanto che sono state abrogate esattamente tutte le norme oggetto del quesito referendario. Conseguentemente vi è una modifica, che abbiamo sottoscritto: nel titolo del decreto-legge vanno sostituite le parole «moratoria nucleare» con le seguenti: «abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari».

per chiedere un chiarimento sostanziale al Governo. Mi rivolgo anche ai colleghi del Gruppo di Italia dei Valori, presentatori degli emendamenti,

differisca di 12 mesi la possibilità di tornare al nucleare. Altrimenti, se avesse avuto la volontà di cambiare rotta, avrebbe non solo espresso parere

5.800 (testo corretto)/105 chiede la soppressione integrale degli articoli 25 e 26 della legge n. 99 del 2009, che è la legge madre da cui originano i decreti legislativi del 2010 e del 2011 che organizzano il ritorno al nucleare. Se si vuole escludere che la ritirata del Governo e della maggioranza sia soltanto soltanto tattica e opportunistica, la via più lineare e trasparente è cancellare per intero la norma da cui sono derivate tutte le norme successive che hanno delineato la *road map* per il ritorno al nucleare in Italia; altrimenti rimane tutto il rischio che questo sia un comportamento ambiguo.

presentatori permettono, vorrei aggiungere la mia firma per sottolineare l'importanza di questa votazione e l'importanza di dire che, se la maggioranza respinge questo emendamento, significa che ha intenzione di proseguire,

decisione da prendere, sulla base della nuova Strategia energetica nazionale, non potrà comunque essere assunta con un provvedimento di rango rango regolamentare, con un decreto del Presidente del Consiglio, o con un decreto ministeriale o interministeriale, ma con norma di legge. Mi pare così evidente! Stiamo abrogando raffiche di norme approvate nell'arco degli ultimi anni, e se il Governo desse il via libera ad una prospettiva di modificazione attraverso provvedimenti di rango inferiore a quello legislativo,

con chiarezza contro questo emendamento del Governo.

perché, come ho potuto dire nel mio precedente intervento, non ritengo che sia un provvedimento giusto. È fatto per altri scopi, e non per quelli che si vogliono far apparire come funzionali all'interesse generale, quindi non può essere condiviso. Non denota neanche eleganza rispetto a due anni e mezzo di vita politica trascorsa nel difendere il programma nucleare, e soprattutto dimostra quanto sia incoerente una politica così ballerina, che imposta un piano energetico con 36 miliardi di euro per quanto riguarda la strategia nucleare e improvvisamente la cancella, senza dare spiegazioni convincenti, se non quelle emotive, che lasciano il tempo che trovano.

e verso anche questo importante settore della ricerca scientifica, quello nucleare. Il mio è pertanto un voto contrario a questo emendamento del Governo. Presidente, l'inganno è disvelato in tutta la sua clamorosa gravità, per cui l'Italia dei Valori vota contro questo emendamento, ed è evidente che porterà

questo un fatto positivo e da sottolineare. Non ci convincono - l'abbiamo detto al Ministro - alcune ambiguità che restano nella stesura di questo emendamento; non ci convince il fatto che non vogliate esplicitamente ritornare a svolgere una discussione nelle Commissioni parlamentari, nelle aule parlamentari, in merito alla strategia energetica successiva. Questi due fatti ci impediscono di esprimere favorevole sull'emendamento in esame. Tuttavia, considerata la portata della decisione che stiamo assumendo, per quanto riguarda Alleanza per l'Italia ed altri colleghi del Gruppo Misto,

motivato che naturalmente chi è contrario al nucleare vedrebbe con favore una decisione del Governo che definitivamente chiudesse questo capitolo. Purtroppo il dibattito e il rigetto di tutti gli emendamenti che potevano rafforzare questa decisione ci mettono fortemente in dubbio su questa volontà. È emerso dal dibattito, dal rigetto di tutti gli emendamenti migliorativi che puntavano sulla decisione definitiva, che il Governo vuole riprendere il nucleare dopo che si siano calmate le acque. Tuttavia, siccome non voglio votare contro un provvedimento che nel cuore vorrei condividere, mi asterrò dal voto.

senatore Ichino, che non è stato di illustrazione di emendamenti, ma piuttosto un intervento in discussione generale. Vorrei soltanto dire che non è contenuta da nessuna parte la strategia difensiva degli investimenti italiani e che la mancanza di attrattività di investimenti esteri non dipende certo, o minimamente, da azioni difensive o

è abbastanza singolare, dopo tutta la discussione che si è svolta, che ci sia un orientamento di totale chiusura rispetto agli emendamenti che sono stati presentati, dopo una discussione - ripeto - che invece è stata molto positiva, sia in Commissione che in Aula. Mi stupisce tra l'altro che non ci sia nessuna forma di approfondimento su un provvedimento come questo che va incontro alle esigenze dell'apparato produttivo italiano, delle piccole e medie imprese. Sarà un argomento che svilupperemo fuori da qui naturalmente.

**Il Senato non approva.** posto ai voti. La discussione che abbiamo fatto precedentemente è terminata, in maniera un po' mesta, con la promessa che faremo una bella conferenza

Noi qui vi proponevamo, invece di dire qualcosa, di fare finalmente qualcosa, cioè Cassa depositi e prestiti, che ha già il controllo di Terna-Rete Elettrica, acquisisce il controllo di SNAM-Rete Gas separandola da ENI; poi fonde le due partecipazioni creando il più grande *player* delle reti a dimensione europea, il quale realizza gli investimenti sulle interconnessioni e, per questa via, fa

produzione di energia nucleare. È chiaro, voi non volete avere una politica energetica a dimensione nazionale ed europea,

tutti fossimo consapevoli di ciò che stiamo votando. Noi chiediamo che il veicolo che assume le partecipazioni nelle società le assuma come partecipazioni di minoranza.

che, se venisse confermata, ci direbbe dove alberga l'ultimo lembo del socialismo di Stato: alberga, purtroppo, in via XX Settembre.

di minoranza e le parole «a condizione che siano caratterizzate da una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e da adeguate prospettive

Grazie,

C'è una ragione, signora Presidente, per la quale questi emendamenti sono identici: è che recepiscono entrambi un punto del parere della Commissione bilancio che aveva valutato opportunamente che queste partecipazioni, che Cassa depositi e prestiti potrà assumere, dovrebbero essere assunte in società che hanno una situazione di equilibrio finanziario e che

che comunque il problema dell'economia italiana è quello di una maggiore internazionalizzazione e non di una chiusura provincialistica, ma questi sono i segnali che noi mandiamo: anziché incrementare i nostri investimenti diretti all'estero, mandiamo il messaggio che una società pubblica, di Stato, può assumere partecipazioni di maggioranza nelle società di diritto comune.

credo che anche questo sia un fatto grave, cioé che tutto quello che abbiamo detto fino ad ora debba avvenire con un decreto di natura non regolamentare

della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Alla fine di tutto questo ci viene regalata una briciola, che naturalmente non possiamo accettare, che stabilisce in maniera un po'

nel definire il decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Il Governo mi pare che non voglia introdurre questo elemento, sicché rimane questa formulazione. Premesso che non sono un esperto di procedure parlamentari, che questa formulazione possa determinare come elemento di procedura il fatto che nel momento in cui il decreto viene trasmesso può essere assegnato alle Commissioni competenti

procedurale che, a mio avviso, è autolesionistico per il Governo, però, poiché siamo in una condizione nella quale si può avere il diritto all'autolesionismo, prendo atto di questo dato, di questo non credo che si possa risolvere il problema con la trasformazione di un emendamento in un ordine del giorno, ritiro gli emendamenti *(Applausi 7.303 e 7.304, perché non è il caso di accedere ad una procedura che è inutilmente paternalistica, ma che non affronta e non risolve i problemi, né quelli politici né quelli parlamentari. *(PD)*. Signora Presidente, il tema che ha posto il senatore Viespoli adesso è affrontato in numerosi emendamenti pressoché di tutti i Gruppi parlamentari,

pareri delle competenti Commissioni parlamentari o della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Hanno presentato emendamenti su questo punto, che è un punto, una norma di buon senso e che quindi dovrebbe essere scontata e che doveva essere contenuta già nel testo, il senatore Viespoli ed altri, il senatore Musso ed altri, il

anche l'emendamento 7.18, e così via. È possibile che il Governo, che pure su questo punto, sottosegretario Giorgetti, si era dimostrato disponibile in Commissione, lo ripeto - a tutelare la dignità, l'autonomia del Parlamento nei confronti di un atto monocratico del Governo su un tema delicatissimo quello dell'acquisizione addirittura di partecipazioni di maggioranza (essendo stato respinto il nostro emendamento) utilizzando il risparmio postale degli italiani, non dimostri un'apertura, un ripensamento?

per carità: avete scelto una strada che è quella delle nazionalizzazioni sul modello venezuelano; va bene. Non capisco però la ragione per la quale non si debba accedere alla tesi che il Parlamento possa confrontarsi con il Governo su quali

il Parlamento; sinceramente non comprendo la ragione per la quale non si debba accedere alla tesi, proposta dai colleghi di maggioranza e di opposizione, che serve solo a fare in modo che il Parlamento e le Commissioni competenti siano consultate e ci sia un confronto sulle scelte strategiche che vengono fatte attraverso attraverso la Cassa depositi e prestiti. Credo che sarebbe anche un modo per definire dei criteri obiettivi e, comunque, mi sembra un'operazione di trasparenza. Sinceramente, stento a comprendere la ragione per la quale non debba essere oggetto di un'approvazione da parte di tutti.

di trasformare in ordine del giorno parte del suo emendamento, quella riguardante il «sentite le competenti Commissioni parlamentari», al di là della polemica sulla questione, abbia delle ragioni, che io sottopongo a tutti.

Il fatto che poi si chieda l'ordine del giorno nasce in questo momento, lo dico in tutta sincerità, da una riflessione, che merita il concreto *iter* di questo provvedimento, su che cosa accada a questo decreto se preventivamente occorre che il Parlamento si esprima - questo non lo riterrei corretto - su una o più società. Potreste capire che timori effettivi

Allora, la proposta di trasformazione in ordine del giorno va in questo senso, cioè quello di impegnare il Governo a considerare esattamente come, sulla base del decreto fatto e trasmesso alle Camere, si possa

dell'accordo alle Camere e la richiesta di un ordine del giorno sul coinvolgimento delle Commissioni parlamentari possa essere una soluzione accettabile.

vada contro gli interessi della Nazione, quelli che, tutto sommato, con questa norma si dice di voler tutelare. La Cassa depositi è prestiti può partecipare a società strategiche scelte da un singolo Ministro

contro ogni logica di libero mercato. Che ne discutano le Commissioni di merito, mi sembra il minimo rispetto a questa impostazione.

sicuramente opportuno un intervento, nelle forme che saranno da valutare; esiste, però, una Commissione che si occupa di questo e che fa una relazione annuale: che la faccia

che vi è lo Statuto della Cassa depositi e prestiti che ha fatto chiarezza su una serie di interventi.

Non vorrei che domani si ripartisse con la compagna referendaria per l'acqua pubblica, che fa scappare gli investimenti all'estero in un settore fondamentale come quello dei servizi pubblici locali.

forse sarebbe bene fare un po' di chiarezza, perché l'intervento del senatore Azzollini rischia di aver seminato un equivoco tra i colleghi, cioè che noi siamo per chiedere un intervento delle Commissioni parlamentari su ogni singola operazione e, quindi, sulle singole imprese che sarebbero oggetto dell'attenzione della Cassa depositi e prestiti. Non è affatto così. Il parere delle Commissioni parlamentari interverrebbe sul decreto che definisce quali caratteristiche debbano avere per strategicità, per ricadute sul sistema economico e occupazionali, le aziende rispetto alle quali la Cassa depositi e prestiti potrebbe esprimere la volontà di un ingresso azionario. Non è un particolare trascurabile, perché, se si perdurasse in questo equivoco, cioè il fatto che staremmo chiedendo che le Commissioni parlamentari si pronuncino su ogni singola operazione, avrebbe pienamente ragione il presidente Azzollini, ma siccome non è così, così, tengo a ribadire che oggetto del voto sarà poi un'altra proposta, quella cioè che le Commissioni parlamentari si pronuncino sulla definizione dei criteri di strategicità, impatto economico e impatto occupazionale dei settori di impresa che possono essere oggetto di intervento da parte della Cassa depositi e prestiti. In questo caso, le Commissioni parlamentari farebbero soltanto il proprio mestiere, senza in alcun modo turbare il mercato, e sarebbero chiamate ad esprimere una valutazione, almeno stavolta, su scelte di politica industriale e finanziaria del Governo. In buona sostanza, il Parlamento non farebbe altro che il proprio mestiere.

La politica deve decidere il perimetro dell'intervento, e su questo sono d'accordo.

Dopo di che agli amministratori della Cassa compete decidere tutto il resto, fare la *due diligence* e verificare l'effettiva ricorrenza delle condizioni per organizzarla. Questa è la visione.

Credo che siamo di fronte allo stesso equivoco che poco fa si perpetuava quando il collega Agostini insisteva sulle differenze tra maggioranza e minoranza, senza rendersi conto che uno può avere anche il 30 per cento ed esercitare il titolo e il diritto di fare, con un patto di sindacato, la maggioranza.

Noi siamo in presenza di uno schema molto chiaro, che prevede un decreto, uno statuto da osservare e i vincoli che all'interpretazione dello statuto hanno dato i soci di maggioranza e minoranza. Gli amministratori sono pertanto obbligati a muoversi lungo i binari delle cose che sono già state decise, che vanno nella direzione di rispettare l'efficienza, la funzionalità e la strategicità dell'intervento. Ai colleghi che insistono per l'altra linea, a sostenere l'importanza del Parlamento, dico che sarebbe fuori dal mondo se noi decidessimo di limitare la capacità del Parlamento di intervenire. Ricordo, però, conclusivamente che la legge istitutiva delle Partecipazioni statali, all'articolo 3, diceva che le imprese dovevano agire secondo criteri di socialità. In funzione di questo e per il concorso delle forze politiche presenti in Parlamento, il modello delle partecipazioni statali ha finito per degenerare, diventando quello che è diventato negli ultimi anni. Credo, invece, che oggi il Governo voglia evitare questa possibilità di degenerazione, lasciando all'autonomia degli amministratori la capacità di decidere cose che riguardano l'operatività delle imprese che si vuole potenziare potenziare e tutelare nella loro italianità. Presidente, colleghi, con questo decreto diamo la possibilità alla Cassa depositi e prestiti di acquisire partecipazioni importanti, come Parmalat, utilizzando il risparmio dei vecchi. Sono nato in un paese, che il senatore Ciarrapico conosce, dove non ci sono sportelli bancari: il paese si chiama Archi, nella Val di Sangro. Non ci sono sportelli bancari, Noi diamo la possibilità di utilizzare il sudato risparmio dei vecchietti, come presumo anche del mio amico senatore De Toni, in Val Camonica, per

con tutto il rispetto per il ministro Tremonti, qui non si tratta di colbertismo: qui mi pare ci troviamo di fronte alla via valtellinese al socialismo. Per questo noi voteremo contro.

l'emendamento 7.8 tenta, ancora una volta, di dare dei criteri all'acquisizione di partecipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti. Vorrei nuovamente ricordare che la Cassa depositi e prestiti gestisce i risparmi dei cittadini, cioè i depositi e i buoni postali, ed è preoccupante pensare che investimenti possano essere fatti solo per criteri dovuti alla politica. Se un deposito garantisce una certa quota di interessi, cosa succede se gli investimenti sottostanti che la Cassa depositi e prestiti effettua non danno remunerazione? Chi garantisce quei depositi? Faccio un esempio che penso possa essere buono per tutti: perché Lactalis? Perché è strategica per il Paese? Non credo. Perché ha dei rendimenti elevati? Forse. Oppure, è un modo per proteggere i produttori di latte leghisti, a scapito dei consumatori?

riguardavano il tema di cui abbiamo dibattuto del parere delle Commissioni parlamentari. Questo emendamento affronta invece il tema del parere della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, che è già istituita per legge, come ha spiegato oggi molto bene la senatrice Bonfrisco, che ha presentato un suo emendamento sulla medesima materia, il

di poter apporre la mia firma all'emendamento 7.311 della senatrice Bonfrisco.

argomento di cui abbiamo discusso fino ad ora, non sarà mai sottoposto al vaglio della Corte dei conti, né del Consiglio di Stato. tutti piena cognizione di che cosa stiamo facendo. Questo decreto non passerà mai né alla Corte dei conti, né al Consiglio di Stato, pur intervenendo su un argomento delicatissimo come l'assunzione di partecipazioni in società, torno a ripetere, di diritto privato. Vorrei che anche i colleghi della maggioranza riflettessero su questo aspetto, perché poi, come è notorio, le maggioranze e i Governi passano.

l'orientamento del Governo e della maggioranza - l'impianto, lo strumentario che il ministro Tremonti si è voluto costruire per farsi un fondo, con il quale poi decide di fatto l'assetto della attività attività imprenditoriale del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo IdV)*. Non ci siamo neppure illusi sulle finalità, perché ci si prende in giro quando si dice che è una norma che serve a contrastare i francesi, quando sappiamo che questi ultimi difendono solo alcuni settori strategici, come la difesa, la sicurezza e

non è altro che la modifica che l'assemblea straordinaria dei soci della Cassa depositi e prestiti ha fatto una settimana fa. Il Parlamento sta ratificando per legge un provvedimento fatto da una

che le persone che costituiranno il consiglio di amministrazione, e quindi il direttore generale e l'amministratore, siano di altissima competenza, comprovata esperienza nel settore e così via, e che la vigilanza sulle caratteristiche sia assegnata alle Commissioni

continuiamo a sostenere con questo emendamento, l'assoluta inopportunità, quanto meno, di utilizzare per queste operazioni il risparmio postale dei cittadini italiani. Che cosa succederà, signor Presidente, signori relatori e signori della maggioranza? Accadrà che un'azienda andrà dal Ministro dell'economia chiedendogli un intervento finanziario sul proprio capitale, al di fuori del controllo del Parlamento e di chiunque altro, e il Ministro dell'economia, per il tramite della Cassa depositi e prestiti (che, come è noto, controlla al 70 disporre liberamente del risparmio postale dei cittadini italiani. È una cosa grave, che non si è mai fatta. L'accoglimento di questo emendamento consentirebbe ugualmente di fare tutto ciò che il Governo e la maggioranza si propongono di fare, ricorrendo però al mercato ricorrendo però al mercato per l'approvvigionamento finanziario e non al risparmio postale, che, fino ad oggi, mai nessuno si

in una fase di crisi sistemica come questa, il risparmio e il sudore della povera gente sono quanto di più sacro ci possa essere. Riflettete bene prima di votare.

o liberali? Al quesito di Totò si possono dare molte risposte, ma francamente non vorrei stuzzicare troppo la maggioranza, che nella stessa giornata è diventata, da liberale,

siano minoritarie e precludano il controllo societario; che sia vietata la partecipazione a patti di sindacato; che quando la Cassa riveste la qualità di socio di minoranza nelle società partecipate, essa è tenuta a presentare una propria lista in occasione della nomina o del rinnovo dell'incarico degli amministratori, ma solo al fine di ottenere l'elezione di un consigliere indipendente, privo di deleghe operative, e di un sindaco della società. Signor Presidente, questo è un emendamento liberale. Spero che la maggioranza non lo bocci, perché sarebbe una scelta particolarmente grave.

procedure di tipo esclusivamente privatistico, mentre nel nostro caso si tratta di uno strumento partecipato al 70 per cento dallo Stato e al 30 per cento dalle fondazioni *ex* bancarie, che ancora non sappiamo se la dottrina interpreti come private o pubbliche), comunque comporta comunque comporta una riflessione e un approfondimento sulla corretta vigilanza, sulle strategie e gli indirizzi. Vorrei rassicurare il senatore Rutelli che non si tratta di politiche industriali né di tipo socialista, né di altro tipo; non si tratta di politica industriale, perché mancano i presupposti e i fondamentali per le politiche industriali nel nostro Paese in questo momento. *(Applausi dal Gruppo PD).* Si tratta piuttosto di uno strumento finanziario che deve poter dare forza e vigore ai processi di crisi finanziaria che dobbiamo superare. Quello che deve preoccuparci non è a quale impresa verrà assegnato questo o quel finanziamento attraverso l'ingresso nel capitale della Cassa, ma l'utilizzo del risparmio postale: 26 milioni di correntisti italiani che portano lì i loro soldi, e quei soldi sono la garanzia degli investimenti della Cassa depositi e prestiti, ma ahimè quei soldi sono garantiti dallo Stato. E se sono garantiti dallo Stato, questo deve poter e saper vigilare attraverso gli strumenti che ha definito in passato. La legge che istituisce la Cassa depositi e prestiti è del 1913; credo che all'alba del 2013 sia il momento di aggiornarla. Accordo volentieri al Governo la mia disponibilità un ordine del giorno, annunciando da adesso la presentazione di un apposito disegno di legge che potrà ritrovare, tra maggioranza e opposizione, le condizioni minime necessarie per aggiornare i poteri della vigilanza. Ringrazio il relatore per il lavoro efficacissimo che ha svolto. Presidente, apprezzo molto la proposta e il ragionamento che ha fatto la senatrice Bonfrisco, ma, quale firmatario dell'emendamento 7.311, non accetto la trasformazione in ordine del giorno. Mi corre l'obbligo di comunicarle il parere della Giunta per il Regolamento, a cui era stato sottoposto tale quesito.

La Giunta per il Regolamento ha così stabilito: «Conformemente alla prassi, quando il proponente ritira un emendamento per trasformarlo in ordine del giorno

dovremmo tentare tutti di uscire, seppur in una fase sostanzialmente elettorale, da una sorta di provincialismo del dibattito e del confronto politico parlamentare che non riesce mai ad individuare un punto di convergenza, neanche quando si tratta di discutere e di affrontare questioni di interesse nazionale.

è parso più concentrarsi sulla dietrologia, su quello che ci poteva essere dietro la scelta del Governo, che sull'importanza di una simile scelta ai fini dell'interesse generale ed ai fini dell'esigenza di collocare finalmente e correttamente il dibattito, non solo senza lasciarlo in bilico tra emotività e sovranità, come inevitabilmente accade e sarebbe accaduto nella vicenda referendaria, ma collocandolo nella dimensione più vasta di carattere europeo. [**Presidenza del entro la quale collocare questioni di tale rilievo. Altrimenti, ci troviamo nella condizione di subordinazione indicata e sottolineata in alcuni interventi, qualche senatore ha evidenziato come siamo stati sostanzialmente noi, con la bolletta energetica nazionale, ad ammortizzare l'investimento delle centrali nucleari in Francia senza

forse nel momento in cui i grandi partiti sono in crisi e in difficoltà: una volta c'era il partito di lotta e di governo, adesso abbiamo il *referendum* di lotta e di governo, cioè il *referendum* che è di lotta per chi intende utilizzarlo come strumento di lotta politica e di governo per chi intende utilizzarlo

tentare di collocare il nostro confronto e il nostro dibattito nel grande scenario che si è aperto, dove noi corriamo il rischio di avere un deficit di presenza politica e di governo. Infatti, dentro lo scenario europeo che si è aperto e dentro dentro la crisi identitaria dell'Europa, dentro l'illusione europea che si potesse costruire l'Europa soltanto sulla moneta unica senza la politica, l'anima, l'appartenenza e l'identità,

un riflusso che va tutto dentro il recupero della dimensione dell'interesse nazionale. Noi abbiamo qualche difficoltà in più, perché non abbiamo questa cultura nazionale, questa narrazione della vicenda nazionale in termini di comunità; non recuperiamo fino in fondo la dimensione fondamentale della politica, politica, e pensiamo che basti un dibattito economico o economicistico per risolvere ed affrontare le questioni ed i problemi che abbiamo di fronte. Non è così. Bisogna dirlo, e lo dico anche per quanto riguarda il dibattito che si è svolto intorno alla vicenda della Cassa depositi e prestiti: non si tratta di interferire, di introdurre elementi di intermediazione della politica, ma di recuperare la politica come capacità di visione,

È importante aver recuperato la funzione di grande interesse dell'area di Pompei come interesse nazionale, seppure poi - diciamoci la verità - sul terreno delle risorse si guardi più al FAS che non alle risorse

aprire. Bisognerebbe recuperare il Sud nella dimensione del confronto e del dibattito, anche perché, sottosegretario Giorgetti, uno dei motivi di perplessità sta nel riferimento all'utilizzo delle risorse postali finalizzate a dare

tra risorse postali e l'intervento a supporto degli investimenti e delle iniziative della Cassa depositi, anche rispetto al rapporto tra Poste e Banca del Sud nella direzione di cui finora si è parlato. Vorremmo riportare ad organicità

altre, altrimenti non riusciamo a comprendere il contesto in cui stiamo operando. Tra dieci giorni dovremo presentare all'Europa il Piano nazionale delle riforme e il Patto di stabilità. Il primo non potrà più essere un elenco di titoli, la solita litania di ritornelli, perché l'Europa richiede il rispetto di alcuni obblighi, tra cui quello della crescita che è divenuta ormai necessaria per la stessa stabilità dei conti. E tutto il nostro Paese si aspetta dopo tre anni di sacrifici risultati concreti. Perché la maggioranza sa bene che anche il venditore più abile, dopo tre anni, se continua a vendere storielle, va in fallimento. È una legge di mercato. Con il Patto di stabilità si pongono alcuni obiettivi rilevanti. Una riduzione del deficit allo 0,2 per cento nei prossimi due anni che, accompagnata a una stima di crescita del PIL ridimensionata ad un modesto 1,1 per cento, significherà che ci dovremo attendere nuove manovre finanziarie che equivalgono a quasi 40 miliardi di euro. La maggioranza e il Governo potranno deciderne i tempi e i modi, a chi fare pagare questa volta il conto, ma stiamo parlando di altri sacrifici veri e pesanti che potranno essere chiesti al Paese soltanto da un Governo che deve avere, prima di tutto, credibilità. Il Ministro dell'economia ha detto che i numeri sono in linea, ma se è lo stesso Ministro che quando va al Sud parla di fiscalità di vantaggio, dopo averla smantellata con i provvedimenti degli ultimi tre anni, e quando va a Milano promette meno tasse con una pressione fiscale in aumento per l'anno prossimo, allora più che di numeri i cittadini hanno bisogno di fatti e di credibilità nel realizzare questi fatti. i fatti contenuti in questo decreto-legge segnano a nostro giudizio, ma non solo al nostro, il fallimento di un Governo. Un Governo - lo abbiamo visto questa mattina - fatto da Ministri e da un Presidente del Consiglio che dicono tutto e il contrario di tutto. Il fallimento di una maggioranza che si tiene insieme soltanto per paura delle elezioni, evocando complotti comunisti e, ancora peggio, il fallimento di una politica economica fatta di continui passi indietro, di scelte smentite dopo pochi mesi, di correzioni del giorno dopo e di improvvisazioni del giorno prima. Andiamo per ordine: il reintegro parziale delle risorse al FUS è la prova provata dell'effetto devastante che i tagli indiscriminati hanno prodotto sulle risorse più importanti del nostro Paese. Per farlo capire, insieme alle opposizioni, si sono dovute sollevare le proteste dei teatri italiani, degli operatori della cultura, delle maestranze delle imprese di settore, a cui si sono aggiunte anche le sollecitazioni del presidente Napolitano per mettere il Governo e questa destra in condizione di non poter difendere l'indifendibile. Solo che a una scelta sbagliata di prima si è posto rimedio con una misura sbagliata di oggi. Giorgetti - un Governo quando soltanto un mese fa il ministro Romani aveva promesso di ridurre di 8 centesimi le attuali accise per riportare il costo della benzina alla media europea, mentre ora sono aumentate di nuovo le accise sul carburante al punto che il prezzo finale è costituito per il 55 per cento da tasse e imposte. Che credibilità possono darvi gli italiani se si sono visti aumentare negli ultimi tempi, mentre vi occupavate di prescrizioni brevi e di processi lunghi, i prezzi degli alimenti e i costi dei consumi energetici? Continuate a portare avanti una politica dei carburanti che non ha nulla di strategico, ma che è diventata uno strumento per risolvere problemi contabili. poi al tardivo programma di intervento per il recupero dell'area di Pompei, è l'epilogo di chi non ha saputo e voluto fare scelte di tutela del nostro patrimonio. Per capirlo ci sono voluti il crollo della "Casa dei gladiatori" e il crollo del ministro Bondi che con le sue dimissioni - lo dico con rispetto umano - si è illuso di immolarsi per il bene della cultura senza capire che è stato la vittima sacrificale di una guerra tutta interna al suo partito e alla sua maggioranza. E come decidono ora di intervenire? Con il pozzo di San Patrizio dei fondi FAS. Per la proroga del divieto di incroci tra stampa e televisione, che ripropone l'eterno conflitto di interessi di un padrone d'azienda che pensa di essere anche il padrone del Paese, per farvi cambiare idea c'è stato bisogno di un altro complotto. Pensate! Sono dovuti intervenire a novembre l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha indicato che la disposizione dei limiti antitrust in una Paese normale è stata concepita proprio a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e informazione. E poi a marzo è dovuta intervenire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha espresso, quantomeno, l'opportunità di sottrarre alle competenze dell'onorevole Berlusconi l'adozione, o la mancata adozione, dell'atto di proroga che toccava direttamente le sue tasche. scelte, signor Sottosegretario, non è contenuto uno straccio di programmazione. La stessa razionalizzazione dello spettro radioelettrico, diciamo la verità sino in fondo, serve al Governo per fare cassa, per mettere in bilancio quei 2 miliardi e 400 milioni di euro che si stima d'incassare dalla vendita di nuove frequenze per la banda larga. Un'asta a frequenze occupate che rischiano di non poter essere assegnate a conclusione della gara (un meccanismo complesso di commissioni, graduatorie regionali, quasi sicuri contenziosi). E lo sanno talmente bene che hanno previsto, nell'eventualità di un insuccesso dell'asta, di fare ricorso, come vuole la legge di stabilità 2011, a nuove riduzioni lineari, a nuove sforbiciate, a nuovi tagli di spesa che andranno a colpire il settore dello sviluppo economico e quello dell'istruzione, della ricerca e dell'università. Per non parlare della cosiddetta moratoria nucleare. L'avevamo definita una presa in giro: ci siamo sbagliati! Ci siamo sbagliati in difetto, però, perché rappresenta una doppia truffa: ai danni dei cittadini e del Paese. Del Paese perché il Governo, dopo tre provvedimenti legislativi sul nucleare, fa marcia indietro, terrorizzato dal crollo di consensi e dai sondaggi, più che dai veri timori degli effetti di una scelta che si rivela per quella che è: ideologica, antieconomica e pericolosa. Berlusconi aveva annunciato che avrebbe posto la prima pietra di una nuova centrale nucleare entro il 2013. Oggi mettete una pietra tombale sulla vostra credibilità e inaffidabilità nella guida del Paese. L'indipendenza energetica del nostro Paese non può essere certo garantita dall'uranio e ora che le Regioni hanno espresso la loro contrarietà a ospitare nuove centrali l'Esecutivo non sa più dove andare a parare e mette su l'alibi della riflessione europea. signor Presidente, mancano i soldi per costruire le centrali nucleari, nessuno le vuole, le scorie radioattive restano per sempre e costa anche mantenerle. Ma è anche una truffa ai danni dei cittadini perché volete manipolare, distrarre, mortificare la regolare espressione della volontà popolare che dovrà esprimersi il 12 e 13 giugno che il Paese non vuole il nucleare e fa soltanto finta di ripensare a una politica energetica che non ha alcuna intenzione di cambiare, come ha confermato nello stesso Documento di economia e finanza testualmente che: «non sono venute meno le ragioni per considerare il nucleare una risorsa utile». utile». La preoccupazione di questo Governo è che gli italiani non dovranno esprimersi, né sul nucleare né, ancora, sui processi che preoccupano il Presidente del Consiglio. Con l'articolo 6, quello sull'Abruzzo, il Governo supera se stesso, passando dalla tassa sulle disgrazie, introdotta con l'ultimo decreto sul federalismo municipale, alle risorse con le disgrazie, perché di questo si tratta. Alle quattro ASL abruzzesi viene data la possibilità di pagare i contratti ai precari con le risorse del decreto n. 39 del 2009 sulla ricostruzione del post-terremoto. Una guerra tra poveri: si tagliano le risorse ai terremotati e le usiamo per i precari. Con l'ultimo articolo poi avete di fatto costruito un fondo che a decidere cosa farne sarà alla fine il Ministro dell'economia, perché non è chiaro chi dovrà decidere realmente, quale italianità strategica vada tutelata, con quali soldi e con quali garanzie.

vera risposta, alla quale questo Parlamento avrebbe dovuto contribuire con il suo dibattito, è quale politica industriale questo Governo abbia intenzione di fare nel nostro Paese. Non l'hanno capito loro, ma il problema è che non l'hanno capito neanche i tanti imprenditori che hanno dichiarato di sentirsi soli. Queste sono le ragioni, signor Presidente, del nostro voto nettamente contrario a questo decreto, con il quale invitiamo anche il 12 e il 13 giugno gli italiani a cambiare il Paese.

materie eterogenee, introduce in sede di conversione degli emendamenti che stravolgono totalmente il testo, a dispetto dei continui moniti del Capo dello Stato e, soprattutto, della qualità e della sostenibilità della nostra produzione normativa. dichiarazione di voto *omnibus*, che cercherò comunque di tenere nei tempi. Articolo 1, sul Fondo unico per lo spettacolo e dintorni. Abbiamo sempre detto, per la verità l'ha detto spesso anche l'ex ministro Bondi, che i tagli lineari, ovunque esiziali, qui mortificavano il settore fino a soffocarlo. Oggi il Governo fa un urgente passo indietro, cancella alcune sue norme, cancella i tagli al FUS, almeno in parte, e cancella l'aumento del biglietto del cinema di un euro. Sia chiaro, non incrementa le risorse per la cultura, come si è sentito dire anche da qualche burlone, ma ripristina in parte quelle che erano state tagliate. Bene il ravvedimento, che però è purtroppo oneroso per tutti i cittadini, famiglie e imprese, attraverso le tasse sulla benzina. Abbiamo già una fiscalità che è al terzo posto in Europa. Andiamo a colpire il settore dell'energia in una fase di ripresa dell'inflazione. Una specie di gioco di prestigio, nel quale alla fine la cultura ha meno soldi, ma la benzina costa comunque di più.

il problema è proprio incidere su quei meccanismi. Questa norma non lo fa. Noi destiniamo già delle risorse che sono, e restano, irrisorie, pari allo 0,18 per cento del PIL, contro il 2-2,5 dei principali Paesi europei, a fronte di un patrimonio culturale che non ha eguali nel mondo. Questa schizofrenia di risorse tagliate linearmente e poi restituite non incide in nulla su quei meccanismi.

essa stessa un grande evento, e straordinarie sarebbero l'ordinaria cura e la manutenzione del nostro patrimonio. L'articolo 3 è un'altra correzione: il cosiddetto milleproroghe attribuiva, con uno svarione o una svista, al Presidente del Consiglio la facoltà di prorogare al 31 dicembre 2011 i termini

L'articolo 4 un passo nella faticosa transizione al digitale terrestre, soprattutto verso una migliore allocazione della risorsa scarsa "spettro radiotelevisivo" fra emittenti televisive e radiofoniche ed operatori delle telecomunicazioni.

e compensazione per le emittenti locali. Così non è stato fatto. Si poteva dare di più del misero 10 per cento del gettito della gara; si potevano favorire aggregazioni di emittenti locali; si poteva evitare di dare come contropartita

norme sulla localizzazione, la realizzazione e l'esercizio di centrali nucleari, abbattendo così un pilastro della piattaforma su cui il centrodestra ha vinto le elezioni. Poi ci sono le domande cattive. Cancella tutti i punti sottoposti al quesito referendario: di fatto, si tratta di una fotocopia del quesito referendario. Quello che i referendari la tragedia di Fukushima ha indotto il Governo a passare da un «avanti tutta» alla moratoria; che cosa è accaduto dopo che lo ha indotto a passare dalla moratoria all'«indietro tutta»? La certezza è un'altra: ora il Paese è senza politica energetica. Continueremo a dipendere dal petrolio e dal gas dei Paesi stranieri; non abbiamo più un progetto di energia nucleare, né un progetto né un investimento sulle energie rinnovabili. Questa è l'insostenibile leggerezza con

vi chiedo quale sia la necessità, in un'economia di mercato retta da un Governo che si dichiara liberale, che un'azienda siffatta sia acquistata dallo Stato. Questa è una norma statalista, che spazza via le residue pretese connotazioni liberali di questo Governo, dopo l'affossamento di tutte le liberalizzazioni Inoltre, è un cavallo di Troia per una nuova infausta stagione di commistione fra politica ed economia e di indebite ingerenze dei partiti nella vita delle aziende. È un passaggio cruciale per il Governo e per la legislatura, e forse anche

l'articolo 2 fa un piano straordinario a "crolli avvenuti"; con l'articolo 3 corregge il suo milleproroghe; con l'articolo 4 di fatto non risolve e confonde ulteriormente il tema del passaggio al digitale; con l'articolo 5 il Governo nega sia la posizione

per emergenze venutesi, guarda caso, a creare, anche se erano ampiamente prevedibili. Sul nucleare un sì, poi un più tardi, poi un no e da ultimo, forse, un non so. so. Per concludere, l'articolo relativo alla Cassa depositi e prestiti segna l'addio definitivo all'impronta liberale, cui si preferisce invece un potere che arbitra l'economia caso per caso. Non è quello che speravamo, non è quello che vogliamo, e dunque voteremo contro questo provvedimento.

tutte le questioni irrisolte, tutti i nodi e le ambiguità contenute nel provvedimento ci impediscono di esprimerci favorevolmente, e però non possiamo non rilevare due questioni,

Allora vediamo i vari articoli. Sul primo, che riguarda il FUS, ci è stato detto che non siamo persone attente alla cultura, che non vogliamo investire nel nostro Paese su questo tema fondamentale. Di fatto, troviamo una risposta seria e concreta, anche se riteniamo che, comunque, la cultura possa trovare nell'attività di partenariato con il privato possibilità di fare interventi importanti. Noi al Nord siamo assolutamente virtuosi da questo punto di vista.

Aumentare il personale a tempo indeterminato senza porre un obiettivo temporale agli interventi fa sì che non si incentivino le buone pratiche di efficienza e di efficacia cui siamo abituati.

che doveva essere un passaggio normativo di cui eravamo convinti. Lo stesso dicasi per la liberalizzazione della banda di frequenza per la messa a gara. sul nucleare, il Governo e il Parlamento testimoniano di essere vicini al Paese, di avere sensibilità e capacità di dialogo con i cittadini e con le associazioni. Non ci meravigliamo e non ci estraniamo da un dialogo che può portare a ripensare e rivedere alcune opinioni. Ci sono fatti mondiali di cui non si potevano segnali premonitori. È giusto che il Governo, come sta facendo, tenga questo collegamento stretto con il popolo e con i cittadini. Per quanto riguarda l'Abruzzo e l'intervento a favore del Servizio sanitario nazionale, testimoniamo una volta di più un atteggiamento di solidarietà e di attenzione a questa terra martoriata da un evento naturale di portata eccezionale.

sentiamo spesso fondi sovrani di altri Paesi intervenire per fare scalate su fondazioni bancarie, su industrie e su altri istituti finanziari; abbiamo sempre ritenuto che l'Italia debba avere una sua leva d'intervento economico-finanziario per quanto riguarda il sistema economico Paese, e quindi possiamo, come ha detto anche il collega Garavaglia, vedere un'attività tipo fondo sovrano. Non ci deve meravigliare.

con senso di responsabilità, stando vicini ai cittadini, rispondendo ai bisogni del nostro Paese. Ce ne assumiamo, ovviamente, come sempre, la responsabilità consapevole. Chiediamo che non ci siano strumentalizzazioni, come quelle che abbiamo sentito, e che si abbandoni quel nervosismo che a volte ho avvertito,

che voteremo tra pochi minuti andrà ricordato perché sicuramente è uno dei capolavori di questo Governo, sia nelle cose positive (poche), che in quelle negative. Sicuramente è il capolavoro delle contraddizioni, di un Governo che ormai non ha più alcuna strategia e che è sempre più lontano dai cittadini e dal Paese. Abbiamo presentato tante proposte. Vittoria Franco, Mauro Agostini, Enrico Morando e altri nostri parlamentari hanno spiegato benissimo la nostra posizione e le nostre proposte, nel merito, nel dettaglio e con grande attenzione, e per questo li ringrazio a nome anche dei cittadini anche dei cittadini italiani, perché prima o poi essi capiranno il lavoro puntuale che abbiamo fatto e comprenderanno la qualità delle nostre proposte. Per la cronaca (se mai se ne occuperà, perché è presa da altri fatti che accadono in Italia: più dalle vicende del Premier che dai problemi del Paese), mi limiterò a riassumere alcune questioni, per cercare di farle capire meglio. La prima questione riguarda la cultura. I beni culturali, il cinema, il grande patrimonio dell'Italia: questa è la materia prima della più grande industria del Paese. Benissimo, questa industria, che era al terzo posto in Europa e anche nel mondo, adesso è precipitata di quattro posti: siamo al settimo posto, e stiamo andando verso l'ottavo. Il turismo del nostro Paese sta precipitando. Bene, qualcuno dirà: «Ma c'eravate anche voi al Governo». Benissimo, degli ultimi dieci anni ci prendiamo il 20 per cento; l'altro 80 per cento però ve lo tenete voi, perché se il turismo oggi precipita ci sarà una piccola responsabilità nostra, ma c'è una grande responsabilità

tagliate il FUS, tagliate nelle soprintendenze, tagliate il cinema, tagliate di tutto, e poi vi accorgete del disastro e cercate di correre ai ripari e di mettere delle toppe.

Ebbene, si torna indietro, si cerca di mettere una toppa, e qual è il provvedimento per dare un po' di risorse alla cultura? accise sulla benzina. Un paio di mesi fa le accise sulla benzina sono state utilizzate per le calamità naturali,

e poi quando vanno a fare la spesa. Se volevate fare una cosa giusta, vi avevamo suggerito di dare una sforbiciatina alle auto blu.

a tutti gratuitamente. È come dire che, se uno ha una casa, essa vale di più, quando la deve vendere, se l'ha affittata. Ma sa benissimo che non la vende, se è affittata.

Dovrete pure capire che in questo modo certificate che siete lontani mille miglia dai problemi del Paese. Se continuate ad andare avanti così,

stop alle rinnovabili. Avete "pastrocchiato" sul risparmio energetico con il 55 per cento. Aumentate le accise sulla benzina. Abbiamo il gas che è il più caro d'Europa.

alla Cassa depositi e prestiti, dove ci sono i soldi dei pensionati. È una di quelle cose che bisogna maneggiare con cura. Se le girate attorno e i pensionati sentono puzza di bruciato, il patrimonio

solo che, votando contro questo provvedimento sembra di essere ai saldi di fine stagione: spero tanto che per voi sia l'ultima stagione.

è chiaro che noi prendiamo l'augurio che questa sia l'ultima stagione come quello che vale sempre, quello scaramantico, che di solito dà luogo a tante nuove stagioni per chi c'è già: e io lo prendo così, da parte del senatore Mercatali. Detto questo, mi avvio ad una rapida e non polemica dichiarazione di voto, esprimendo le ragioni per cui il Popolo della Libertà convintamente voterà a favore del provvedimento in esame. Mi soffermerò

ma il dato che connota questo decreto‑legge è che, per la prima volta, un bene dello Stato, come le radiofrequenze, viene concesso non gratuitamente.

un regolare bando e un'importante previsione di incassi, che noi speriamo possa essere conseguita e realizzata. Certo, il problema è esattamente questo, ma di questo - ripeto - abbiamo discusso attentamente. Ci sono dei problemi che vengono appunto dalla concessione gratuita delle radiofrequenze che fu fatta in altri periodi, ma è meglio non discuterne qui. Oggi

Speriamo che porti al risultato sperato, per evitare quella altrettanto corretta e incisiva copertura che è stata prevista come salvaguardia. Come noto, sono stati già operati gli accantonamenti per l'eventuale e malaugurato l'eventuale e malaugurato insuccesso dell'asta: un modo trasparente e serio, che espone il Governo alle critiche politiche (come è giusto che sia), ma che è stato fatto con puntualità. Quindi, c'è una buona copertura, e per la prima volta finalmente, un bene dello Stato con una regolare asta, un bando e a un certo prezzo, che noi ci auguriamo sia il più alto possibile. La seconda questione è quella del nucleare. La polemica

anzi - il Governo ottempera a quella previsione del legislatore, che era la previsione corrente: se i cittadini chiedono un *referendum*, il modo normale per rispondere a quell'esigenza è fare una legge che vada incontro. Noi lo abbiamo fatto. Capisco bene - mi consentirete solo una parte di piccola e simpatica polemica - che quando

un Governo prenda atto di una situazione che ha modificato radicalmente la percezione del nucleare e cambi radicalmente il suo programma. Lo fa con questo intendimento, per un rispetto straordinario. Il

volontà più distesa dell'intera popolazione. Quindi, mi pare una norma seria, fatta bene, che nasce da motivazioni profonde e che tra l'altro vi sorpassa. Pazienza: abbiamo fatto bene. Per la Cassa depositi e prestiti, anche in questo

Innanzitutto, voglio ricordare a tutti che il capitalismo è cambiato profondamente. I fondi sovrani, ossia qualcosa che nemmeno era immaginabile fino a pochi anni fa, oggi sono delle forze finanziarie spaventose, tali da poter comprare il debito di un Paese europeo intero senza colpo ferire e tanto da essere addirittura il forziere dei titoli di Stato della più grande economia mondiale. Agiscono addirittura in questo modo, e quindi bisogna che uno Stato si attrezzi a queste enormi novità. Questo vale per i fondi sovrani; questo vale per il fondo salva-Stati dell'Europa, che risponde in qualche modo alle esigenze e si attrezza in questo senso. c'è una specificità italiana dalla quale nasce l'articolo 7 ed è quella di una situazione nella quale - diciamoci la verità alcuni provvedimenti elaborati sia dai Governi di centrosinistra che da quelli di centrodestra, che io condividevo (per esempio quello volto ad aiutare la ricapitalizzazione delle imprese, che è un problema serio in Italia) non hanno avuto i risultati che avevamo sperato. Abbiamo ancora molte imprese sottocapitalizzate, che per ciò stesso possono essere preda non soltanto di normali meccanismi di mercato, ma anche di tentativi di spostare i centri di comando delle grandi imprese multinazionali, con un evidente

e noi abbiamo colto tale esigenza. Abbiamo un sistema industriale vivacissimo, sottocapitalizzato; abbiamo anche un problema di ricapitalizzazione degli istituti di credito. Quelli italiani sono sicuramente migliori, ma hanno bisogno di ricapitalizzazione per Basilea 3, e lo Stato attinge ad una grande risorsa, ossia la Cassa depositi e prestiti, e la rende funzionale.

signor Presidente, il Senato ha lavorato benissimo, mantenendo integri, secondo le sue precise indicazioni, gli argomenti che il Governo ci aveva posto e facendo in modo, in questo caso, che il decreto rimanesse intatto

passare al voto finale, vorrei cogliere l'occasione per indirizzare a voi e ai vostri familiari i miei migliori auguri di buona Pasqua.